interno si colloca un'azione volta al contrasto al terrorismo, anche alla luce della crescita e della diversificazione della minaccia terroristica nella regione dell'Africa occidentale. Del resto, come il recente attentato di Dacca ci ha confermato, il jihadismo ha ampliato la sua caratura geografica, dall'Africa all'Asia, incuneandosi proprio in quelle società dove problemi politici e sociali, veri e propri fallimenti degli Stati e problemi persistenti nella costruzione statuale hanno radicato la follia del terrorismo di matrice islamica. un fenomeno che continua a colpire barbaramente civili inermi in varie parti del mondo. Nella consapevolezza dell'interdipendenza tra sicurezza e sviluppo, da parte italiana ed europea si tende sempre più ad adottare un approccio integrato, che includa gli aspetti sociali e quelli di carattere umanitario e di contrasto al terrorismo. Come affermato dal ministro Gentiloni alla Camera dei deputati il 13 luglio scorso, la prospettiva dell'Africa rappresenta una delle sfide più importanti che l'Italia e l'Europa si trovano davanti. In questo ambito, il nostro Paese, al di là delle dichiarazioni rituali che da tempo si pronunciano sull'Africa, sta svolgendo un ruolo di primo piano, riportando il continente africano in cima all'agenda politica, anche con azioni a livello europeo.

Sin dall'esercizio da parte del nostro Paese della Presidenza dell'Unione europea ci siamo occupati della promozione della cooperazione allo sviluppo in una prospettiva di lungo periodo. In tale ambito, oltre ai ben noti processi di Rabat e Khartoum, volti a promuovere una gestione comune fra Europa e Africa del fenomeno migratorio, uno strumento fondamentale è rappresentato dal «Fondo europeo di emergenza per affrontare le radici del fenomeno delle migrazioni illegali in Africa», adottato a La Valletta nel dicembre 2015. Come dicevo, il Governo italiano in questa ambizione e visione per il continente europeo si è fatto recentemente promotore del *migration compact*. L'approccio italiano è stato recepito nella Comunicazione nella Comunicazione della Commissione europea dello scorso 7 giugno sulla definizione di un nuovo quadro di partenariato, a cui il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno ha dato un forte sostegno politico. Si tratta adesso di elaborare e finanziare accordi *ad hoc* hoc* per i Paesi prioritari (Nigeria, Niger, Etiopia, Senegal, Mali) collegati ai flussi migratori lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Per quanto concerne un rapporto tra migrazione e terrorismo, è ovvio che non c'è un nesso causale, ma è evidente che i flussi migratori da quei Paesi sono anche frutto di un'instabilità e di un pericolo per le popolazioni in oggetto. Non a caso, per quanto concerne la Nigeria, il Governo italiano segue con grande attenzione l'evoluzione della situazione sul terreno, dove permane una forte insicurezza nonostante la liberazione di gran parte dei territori occupati da Boko Haram. Al momento, si stima siano ancora in mano ai guerriglieri circa 360 tra 360 tra studentesse, donne e giovani uomini, in gran parte rapiti tra aprile e giugno 2014 nello Stato del Borno. Il Governo nigeriano ha confermato le difficoltà nel rintracciare le studentesse rapite, molte delle quali vendute come mogli nei paesi della regione o costrette a sposarsi ai terroristi, anche se rimane la speranza di ritrovarle con la progressiva riconquista dei territori occupati dai terroristi. L'Italia e l'intera comunità internazionale, compresi i Paesi africani vicini che partecipano alle operazioni di liberazione di queste regioni, hanno sin dal principio fermamente condannato l'episodio di Chibok, emblematico della volontà dei terroristi di impedire con tutti i mezzi l'emancipazione femminile e, più in generale, il progresso sociale della popolazione.

l'iniziativa nigeriana di inserire Boko Haram nelle liste delle organizzazioni terroristiche legate ad Al-Qaeda e sostenendo la concertazione internazionale per combattere il fenomeno del terrorismo islamico in Nigeria, messa in atto fin dal 2014. In tal modo, è stata favorita una mobilitazione regionale regionale contro il terrorismo, prevedendo lo scambio di informazioni e l'istituzione di pattuglie coordinate, tra cui la Multinational joint task force (MNJTF), costituita da Nigeria, Ciad, Niger, Benin e Camerun per contrastare le azioni di Boko Haram nel bacino del lago Ciad. Anche grazie all'impulso e al sostegno di tutti i Paesi europei e dell'Italia, proprio l'Unione europea ha messo a disposizione della costituenda forza internazionale un contributo di 50 milioni di euro ed è intervenuta a sostegno delle forze di sicurezza africane attraverso l'invio di esperti di sicurezza, fornendo il proprio contributo anche nel campo della riforma della giustizia penale e dell'assistenza umanitaria (acqua e sanità). Oltre a ciò, l'Italia ha realizzato alcuni progetti nel settore della formazione in favore delle forze di sicurezza nigeriane, quale ulteriore contributo italiano alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata in Nigeria. Quanto alle iniziative sul piano umanitario, l'Italia partecipa attivamente alle discussioni in corso a livello di capitali europee nell'ambito del gruppo aiuti umanitari dell'Unione europea. Inoltre, la cooperazione italiana ha erogato direttamente nel marzo 2015 un contributo di emergenza di 350.000 euro per sostenere le attività di di assistenza a sfollati interni e comunità ospitanti nel Nord del Camerun colpiti da Boko Haram. Vorrei pertanto concludere confermando il forte impegno dell'Italia in una visione strategica di riapertura di un rapporto tra Europa ed Africa, al di fuori dei rituali progetti di cooperazione o di condivisione e di solidarietà, costruendo su iniziative concrete un sostegno alla crescita di un Paese che, tra flussi migratori, problemi persistenti di povertà e nuovo radicamento di forze legate al jihadismo (prima di Al-Qaeda e adesso del califfato di Daesh) mettono in serio pericolo la vita di tanti cittadini costretti a fuggire. Le crisi e le sfide in materia di sicurezza in Africa, con particolare riferimento al fenomeno di Boko Haram, costituiranno peraltro una delle principali priorità del nostro Paese e del Parlamento

che, come lei ha avuto modo di vedere, anche in relazione ai fatti ascritti, sono purtroppo contemporanee; anzi, per alcuni aspetti sono una prima una prima evidenza, in particolare in relazione ai Paesi colpiti che lei ha citato. Naturalmente ci riferiamo alla Nigeria, ma anche al Camerun, al Mali, al Ciad, eccetera; tutti Paesi che hanno visto una progressione verso la violenza e l'occupazione da parte delle forze che si sono richiamate ad al-Baghdadi e allo stesso Stato islamico e che hanno reso ancora più difficile, se possibile fino

valutate con difficoltà nelle varie istituzioni e nei vari tribunali chiamati a vagliare quelle posizioni, proprio perché è difficile determinare le ragioni profonde della partenza, mescolandosi ragioni diverse. Da una parte certamente c'è l'occupazione di forze fortemente violente e che limitano le libertà individuali, rendendole, com'è evidente, in molti casi impossibili; dall'altra

a mettere insieme le questioni, cercando di non vederle l'una staccata dall'altra. Lei ha parlato prima della cooperazione, della *partnership* e del nostro intervento in ambito internazionale, volto non soltanto ad aiutare le popolazioni di queste realtà africane, ma anche a rafforzare la loro capacità la loro capacità di difesa interna e di sostenersi con adeguatezza dal punto di vista scolastico ed istruttivo. La prima interrogazione nasceva proprio dal rapimento di oltre duecento ragazze da parte di Boko Haram. significativo il fatto che fossero più di duecento queste studentesse di una scuola superiore e che fosse perciò in evidenza la loro emancipazione, come donne e come soggetti civili della Nigeria, quindi capaci di promuovere una società diversa per il loro futuro. Purtroppo ad oggi ancora non sappiamo quasi nulla Questo ci dice quindi come la battaglia sia su più fronti: sul fronte educativo e dell'istruzione, sul fronte della cooperazione internazionale e degli aiuti umanitari, ma anche sul fronte della pace e dell'aiuto ad una difesa interna ed anche

quei territori. Questo è l'auspicio e la ringrazio per queste informazioni ulteriori che, in qualche modo, portano in evidenza la grande volontà, che da questo Governo non è mai venuta meno sin dal momento in cui è entrato in carica, di promuovere una forte cooperazione internazionale. C'è, d'altra una volontà di procedere insistendo, anche nelle sedi internazionali opportune (e credo che sia importante ciò che si può fare in quegli ambiti), per promuovere la pace, la cooperazione e soprattutto la libertà di questi popoli sottomessi a condizioni inaccettabili. La ringrazio davvero.

Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Pepe chiede di conoscere quali siano state le motivazioni alla base del sequestro di sciarpe e di una decina di bandiere con lo stemma del Regno delle Due Sicilie, che sarebbe stato operato da personale della Polizia di Stato in occasione della partita di Europa League del Napoli, tenutasi presso lo stadio San Paolo il 5 novembre dell'anno scorso. Ciò in un contesto che vede impunite negli stadi di tutta Italia l'esposizione di simboli e striscioni e la diffusione di cori con contenuti razzisti e intolleranti. Evidenzio in via preliminare che in occasione del predetto incontro di calcio, non è stato eseguito alcun sequestro di sciarpe o di bandiere recanti lo stemma delle Due Sicilie. Inoltre non si ha riscontro, dalle notizie acquisite, né dell'adozione di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, il cosiddetto DASPO, né dell'esecuzione di arresti nei confronti di coloro che si rifiutavano di consegnare i vessilli in questione. Su un piano più generale, rappresento che da tempo questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi quello di garantire il regolare e sereno svolgimento delle competizioni calcistiche, impedendo che esse possano costituire l'occasione per manifestare ideologie che nulla hanno a che vedere con l'agonismo sportivo. A tal fine, opera l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha il compito di assicurare, attraverso apposite linee guida, l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale delle disposizioni e delle misure di prevenzione e contrasto di incidenti e turbative in occasione delle competizioni sportive. In particolare, l'Osservatorio ha previsto, già dal 2007, il divieto di introdurre vessilli e bandiere all'interno degli impianti sportivi, ad eccezione di quelli riportanti i colori della propria squadra e degli Stati rappresentati in campo. L'introduzione negli impianti di simboli non pertinenti all'evento in programma è subordinata all'autorizzazione del Gruppo operativo di sicurezza, appositamente costituito dal citato Osservatorio, nel rispetto della normativa vigente. Analoga autorizzazione è prescritta in ogni caso per l'introduzione negli stadi di mezzi di diffusione sonora. Ciò al fine di assicurare sia la qualità dello spettacolo, che verrebbe pregiudicata dall'esposizione di messaggi contrari al buon gusto e all'etica sportiva, sia la sicurezza degli spettatori, atleti e quanti siano interessati alla gestione dell'evento sportivo. In ordine all'asserita impunità di cui godrebbero, negli stadi italiani, gli autori di gesti o messaggi d'intolleranza o dal contenuto razzista, assicuro ovviamente che l'Amministrazione dell'interno è fortemente impegnata anche su questo aspetto. Il citato Osservatorio, attraverso numerose determinazioni, ha fornito indicazioni finalizzate a far rispettare il divieto di esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o di intolleranza attraverso la diffusione di cori o l'esposizione di scritte all'interno degli impianti sportivi e nell'area esterna ad essi riservata. Tale impegno è attestato anche dall'attività della *task force* per la sicurezza delle manifestazioni sportive, istituita all'inizio del 2014 con la partecipazione di tutti gli attori del mondo del calcio, per individuare e analizzare nel dettaglio formule innovative mirate al miglioramento dei livelli di sicurezza negli stadi italiani. In attuazione del pacchetto delle misure di sicurezza varato da tale organismo il 7 aprile 2014, sono state avviate iniziative finalizzate a realizzare nuove campagne di prevenzione delle varie forme di discriminazione, da adottare negli impianti sportivi anche in collaborazione con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Concludo, evidenziando che l'obiettivo che il Governo, in stretto raccordo con le società sportive, intende perseguire con il complesso delle misure che ho appena descritto è quello di restituire lo spettacolo calcistico ad una dimensione di normalità e serenità che invogli anche ad una maggiore frequentazione dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive da parte delle famiglie e delle persone di giovane età.

sappiamo chi è stato ma comunque qualche problema l'abbiamo avuto) è entrata a far parte delle simbologie associate alla squadra del Napoli calcio e soprattutto alla città e a quel Sud Italia inteso come erede culturale del glorioso Regno delle Due Sicilie con una valenza storica e culturale più che politica. Non è questione marginale, perché sta generando un crescente risentimento. Mi creda, non è una questione da niente, non è una questione irrilevante, è una questione di identità,

valori in cui si riconoscono migliaia di cittadini, con orgoglio, appunto, ma senza negare la Repubblica e lo Stato. È una bandiera che rappresenta le nostre radici,

con l'interrogazione all'ordine del giorno viene richiamata l'attenzione del Ministro dell'interno sulla manifestazione che, come già lei ricordava, ogni anno, il 25 aprile, militanti di destra promuovono ad Aprilia, per ricordare i caduti di un battaglione della X flottiglia MAS. In relazione alla rievocazione di quest'anno, il senatore Cervellini ha chiesto un intervento del prefetto di Latina volto ad evitare che l'evento si svolgesse ancora una volta in concomitanza con le celebrazioni della liberazione dal nazifascismo. Ovviamente, la mia sarà una risposta a consuntivo, che darà conto dell'attività svolta dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza e dalle forze di polizia per prevenire turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Effettivamente da svariati anni, la mattina del 25 aprile, alcuni militanti di destra sono soliti radunarsi nella frazione Campoverde di Aprilia, davanti al cippo commemorativo dei caduti della Repubblica sociale italiana, per sostarvi per alcuni minuti, depositare una corona di fiori e, a cerimonia conclusa, recarsi a Nettuno presso il cimitero dedicato ai caduti della Repubblica sociale italiana. Negli ultimi anni, e precisamente a decorrere dal 2013, in coincidenza con il raduno si svolge una mobilitazione di opposto segno politico, con momenti di tensione controllati dalle forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Quest'anno, in vista del 25 aprile, sia il dirigente nazionale del movimento politico La Destra sia il presidente dell'Associazione nazionale partigiani di Aprilia hanno presentato in questura un regolare preavviso di manifestazione. Nei giorni successivi non sono mancate esternazioni ingiuriose e intimidatorie nei confronti dell'ANPI da parte di un esponente di vertice del gruppo estremistico di destra denominato Militia; esternazioni peraltro pubblicamente disapprovate da esponenti del movimento di destra promotore della commemorazione. La questione è stata oggetto di esame nel corso di una riunione di coordinamento delle forze di polizia, convocata dal prefetto di Latina il 13 aprile. L'analisi svolta ha evidenziato come non sussistessero controindicazioni alle due riunioni e come, in realtà, gli unici aspetti di criticità riguardassero il loro concomitante svolgimento. In ragione di ciò, le autorità di pubblica sicurezza hanno adottato tutte le misure e i dispositivi idonei a prevenire turbative dell'ordine pubblico, imponendo anche speciali prescrizioni volte giustappunto a evitare la simultaneità dei raduni. Alla commemorazione organizzata dai movimenti di destra hanno partecipato circa 100 persone, tra le quali diverse decine di militanti dei gruppi Militia e Forza nuova. Contestualmente, nel piazzale antistante, si sono radunate, in netto anticipo rispetto all'orario prescritto dalla questura, circa 40 aderenti all'ANPI e rappresentanti dei movimenti di sinistra che hanno scandito *slogan* antifascisti. Tra i contromanifestanti è stata notata la presenza anche del senatore interrogante. La cerimonia si è svolta senza interruzioni e il dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto per l'occasione ha evitato che si registrassero momenti di tensione. Questi i fatti, dai quali emerge come il prefetto e il questore di Latina, garantendo lo svolgimento di entrambe le manifestazioni in un'adeguata cornice di sicurezza, abbiano realizzato un equo contemperamento dei vari interessi giuridicamente rilevanti in gioco e, così operando, si siano mossi nel solco dei principi costituzionali e delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che delimitano i poteri delle pubbliche autorità in occasione dell'indizione di manifestazioni pubbliche.

Il punto che si pone è l'inaudita autorizzazione a iniziative che vedono la celebrazione pubblica e ostentata, con il ricorso anche

in occasione del Secondo conflitto mondiale e che faceva dire al prefetto di Milano dell'epoca, nel 1944, che era una realtà che andava allontanata dalla città. In quei luoghi e poi nella ritirata successiva, nel Centro e nel Nord d'Italia, sono proseguiti da parte degli esponenti di questo battaglione, crimini, persecuzioni, rappresaglie e altri misfatti odiosi.

Abbiamo a cuore il ricordo, quando è ricordo - quindi senza ostentazione e senza manifestazioni pubbliche - nei luoghi dove i ricordi privati devono essere e soprattutto non il giorno del 25 aprile, che non è la festa di una parte, ma la festa del popolo italiano, che attraverso la lotta di liberazione ha determinato questa democrazia e questa Costituzione democratica antifascista.

senatori, i fatti accaduti il 29 giugno scorso a Sesto Fiorentino, in occasione di controlli di *routine* effettuati su un'azienda cinese da personale dell'ASL, in collaborazione con operatori di polizia, si sono caratterizzati per la reazione violenta e intollerante alle verifiche in corso, ritenute vessatorie e discriminatorie. L'intervento delle Forze dell'ordine, improntato all'equilibrio e a una accorta gestione dei momenti di maggiore tensione, è riuscito a riportare la calma tra i manifestanti, mentre l'attività svolta da questura e prefettura di Firenze è servita a scongiurare che altri episodi di protesta potessero essere inscenati nelle giornate seguenti. In questa cornice, assai utile è stato anche il rapporto di collaborazione instauratosi con le autorità consolari cinesi, con le quali è stato sempre attivo un canale di dialogo grazie al quale sono stati fugati ingiustificati sospetti circa le motivazioni effettive dei controlli. In ogni caso, i disordini in questione sono tuttora oggetto di attività investigativa da parte delle squadre mobili di Firenze e Prato, nell'ambito di un procedimento penale instaurato presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze. In realtà, è dal 2014, a seguito dell'incendio di un capannone a Prato nel quale persero la vita sette cittadini cinesi, che nel distretto manifatturiero toscano, in particolare dell'area Firenze-Prato-Pistoia, viene attuato un piano straordinario triennale di controlli, eseguito con cadenza mensile e basato su verifiche a tutto tondo. Non è, infatti, solo l'aspetto commerciale che viene posto sotto osservazione, specie per il profilo della contraffazione dei marchi, ma anche quello della prevenzione del fenomeno del lavoro nero, di quello irregolare e sommerso, della protezione sociale dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Naturalmente, si tratta di controlli indirizzati verso qualunque attività imprenditoriale, indipendentemente dalla nazionalità del gestore o delle maestranze, il cui principale scopo è far sì che vengano rispettate rigorosamente le regole della corretta corretta competitività, a beneficio del mercato e degli stessi lavoratori, nonché - c'è da aggiungere - ad evitare che si ripetano episodi come quelli appena citati. Questa attività, che seleziona preventivamente la tipologia di aziende da sottoporre a controllo, si basa su periodiche ispezioni degli uffici territoriali del Ministero del lavoro, nonché su accessi effettuati da tecnici delle competenti ASL. In entrambi i casi, le verifiche si giovano dell'apporto collaborativo di operatori di polizia, dando luogo talora a veri e propri accessi congiunti. Il metodo di lavoro finora attuato ha dato positivi risultati, consentendo di far emergere consistenti sacche di irregolarità nel bacino di Firenze-Prato-Pistoia, dove gli operatori ASL hanno controllato, tra settembre 2014 e maggio 2016, 5.823 aziende, il 64 per cento delle quali ha palesato carenze o criticità di vario tipo e gravità. È significativo che l'esame del *trend* nel tempo di tali controlli abbia evidenziato un progressivo miglioramento delle percentuali delle aziende risultate in regola, a testimonianza della validità dell'approccio adottato dalle pubbliche autorità. Sul fronte del contrasto al lavoro nero, appaiono rilevanti anche i dati relativi alle attività delle direzioni territoriali del lavoro di Firenze e di Prato, che hanno effettuato, nel corso del 2015, per entrambe le Province, circa 4.000 accessi ispettivi. All'esito di queste ispezioni, sono state inflitte numerose maxisanzioni per lavoro nero e per impiego di manodopera clandestina. Quanto ai profili di criminalità economica e al reinvestimento e riciclaggio dei profitti illeciti, provenienti anche da elusione o evasione fiscale, riferisco che, tra il 2014 e il 2016, i reparti della Guardia di finanza hanno effettuato, nelle sole Province di Firenze e Prato, 776 interventi ispettivi nei confronti di ditte individuali e società riconducibili a soggetti di etnia cinese. Tali attività hanno permesso di: di: individuare complessivamente 173 evasori totali o paratotali; proporre il recupero a tassazione di una maggiore base imponibile lorda pari a circa 248 milioni di euro; euro; constatare ricavi non contabilizzati per circa 8 milioni di euro e un'evasione dell'imposta sul valore aggiunto per oltre 57 milioni di euro. Severo è stato anche il contrasto ai *money transfer*, che ha consentito di accertare, sul fronte della circolazione transfrontaliera di capitali, importi non dichiarati per circa 21 milioni di euro nei confronti di oltre 2.000 soggetti di nazionalità cinese che hanno operato nell'intero territorio nazionale. Nei settori dei prodotti contraffatti e di contrabbando, la Guardia di finanza ha accertato, nell'arco di un biennio, violazioni connesse alla falsa denominazione d'origine e alla pericolosità per la salute dei consumatori, nei confronti di 2.348 cittadini cinesi, sottoponendo a sequestro quasi 90 milioni di prodotti irregolari in tutto il territorio nazionale. Più in generale, assicuro che le autorità provinciali di pubblica sicurezza e le forze di polizia continueranno a mantenere alta l'attenzione sui traffici, sulle forme di sfruttamento e sulle attività illecite di varia natura all'interno delle comunità cinesi, al fine di cogliere segnali premonitori e accadimenti che rendano necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione o contrasto dei fenomeni criminosi. Rispondendo, infine, alla specifica sollecitazione riguardante l'associazione cinese denominata Cervo bianco, informo che, in base alle risultanze attuali delle indagini, la medesima risulta coinvolta nei fatti di Sesto Fiorentino solo in via marginale e a scontri già iniziati. La squadra mobile di Prato ha accertato, infatti, che alcuni dei componenti dell'associazione si sono mossi da Prato per recarsi a Firenze solo in tarda serata, chiamati a raccolta da una convocazione basata sul passaparola, avvenuta tramite *chat* telefoniche in uso agli appartenenti alla medesima Tuttavia, sono ancora in corso attività investigative finalizzate a comprendere l'effettiva consistenza e portata della partecipazione dell'associazione ai disordini di cui abbiamo parlato. Come riportato nell'interrogazione, la mattina del 1° luglio, la squadra mobile di Prato, indipendentemente dai fatti di Sesto Fiorentino, aveva già in programma lo svolgimento di perquisizioni a carico di sette componenti e delle due sedi dell'associazione. Le ipotesi di reato contestate e che hanno portato alle perquisizioni riguardano l'associazione a delinquere finalizzata ad atti di violenza per motivi etnici e con finalità razziste. Per quanto emerso nel corso delle indagini, il gruppo delle persone perquisite aveva organizzato e portato a termine ronde e *raid* punitivi ai danni di soggetti di etnia maghrebina, accusati di compiere rapine in danno di cittadini cinesi. Nel corso delle perquisizioni sono state identificate diverse persone con precedenti per immigrazione clandestina e altri reati e sono stati sequestrati oggetti utilizzati impropriamente, come mazze per colpire le potenziali vittime. Uno dei componenti dell'associazione, un detenuto in semilibertà per omicidio, è stato riconosciuto come uno dei cittadini cinesi che la sera del 29 giugno erano presenti a Sesto Fiorentino e poi, il 30 giugno, manifestavano di fronte al tribunale del capoluogo della medesima città, in occasione del rito per direttissima a carico dei cinesi arrestati la sera precedente. A tale soggetto è stata ovviamente revocata la semilibertà.

proprio i dati che lei ha riferito mostrano in tutta la sua gravità un fenomeno pervasivo di illegalità e le responsabilità anche dal suo Dicastero per il fatto che questa situazione si sia venuta consolidando negli anni. due aziende su tre si rivelano irregolari, noi abbiamo chiaro che servono misure straordinarie a repressione di questo fenomeno, misure straordinarie che ancora non vediamo, eppure da mesi sto denunciando questa situazione e proponendo dei correttivi alla vostra attenzione: ad esempio, nella mia interrogazione del 28 aprile scorso ho rivolto al Governo

Per anni ci avete detto che la Cina sarebbe stata il mercato del futuro per le imprese italiane, che le nostre merci avrebbero trovato nuovi sbocchi presso l'emergente classe media cinese, che l'entrata della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio era il più grande affare della storia; dopo quindici anni, però, scopriamo ma lo sappiamo da tempo - che la nostra bilancia commerciale mostra una Caporetto: siamo il terzo Paese con il più alto *deficit* commerciale verso la Cina, siamo noi a essere invasi dalle loro merci. L'unico Paese europeo a essere in attivo è la Germania. Per le nostre imprese, che hanno una vocazione manifatturiera, è un disastro. L'Italia è di fatto il *terminal* di una nuova via della seta, che loro chiamano *one belt, one road*: un'enorme infrastruttura che parte dalla Cina, via Cina, via ferroviaria e marittima; attraversa sessanta Paesi e coinvolge 4 miliardi di persone, ed è lo sfogo essenziale per la sovracapacità produttiva della Cina e di tutto il Sud-Est asiatico. La Cina ha un regime statalista e autoritario ma lungimirante, e ha costruito da molti anni le sue basi in Italia. Prato, Milano, Padova sono le teste di ponte consolidatesi negli anni, malgrado i ripetuti scandali per le violazioni sulle norme del lavoro, sul commercio di prodotti contraffatti e nocivi e sugli enormi spostamenti di denaro sospetto attraverso i *money transfer*: proprio quelli che lei ricordava. Sembra che lo scopriamo oggi, ma un sistema di questo tipo non si improvvisa tipo non si improvvisa e nasce dall'illegalità e dal vantaggio competitivo che garantisce quelle imprese, ma si consolida grazie allo storico e ininterrotto *laissez faire* della sinistra che governa quei territori. Lei ci riporta l'esempio del tragico incendio

la municipalizzata locale è andata a perlustrare quei capannoni, ma si è limitata a censire la metratura dei dormitori all'unico scopo di ricavarne la fiscalità, cioè le tasse sull'asporto rifiuti. Tutto normale. Eppure, le cose si sapevano e venivano denunciate dai nostri imprenditori, secondo i quali, se un appartamento ha svariati kilowatt di fornitura elettrica, non è un'abitazione ma un laboratorio; se trovo dieci macchine da cucire e solo due operai regolari, quello è un luogo di illegalità e di elusione. Ci chiedono di consentire alle nostre Forze dell'ordine - qui, Sottosegretario, è la responsabilità sua o del suo Dicastero - di fare i controlli di notte, perché di notte i nostri imprenditori dormono, poco, e lavorano di giorno, mentre il contrario succede invece in molte, troppe imprese cinesi. Allora dobbiamo decidere cosa vogliamo fare, perché abbiamo concesso una sorta di extraterritorialità in cui le imprese cinesi hanno una sostanziale impunità Toscana, territorio roccaforte della sinistra, ma forse potremmo dire, più precisamente, feudo incontrastato del nostro Presidente del Consiglio e delle sue sodali stampelle di Governo.

dove regna l'illegalità, dove c'è addirittura una sorta di polizia privata che, ancorché marginalmente, interviene in fatti gravissimi, dove un controllo delle autorità sanitarie viene ostacolato con la forza. Non possiamo minimizzare questi segnali, perché ci dicono che quella che nasce come illegalità sul piano commerciale e fiscale è diventata un qualcosa di gravissimo sul piano dell'ordine pubblico. È questa la punta dell'*iceberg* che non si riesce a ricondurre all'enorme sommerso che sta sotto. Abbiamo bisogno di normative straordinarie e urgenti. Se questo è il sistema economico che ha in mente il presidente del Consiglio Renzi, noi non possiamo permettere che ci venga a toccare nella nostra sicurezza e

in riferimento all'interrogazione in oggetto relativa alle peculiarità del bacino del fiume Reno, e in particolare alle criticità spondali connesse prevalentemente a fenomeni di erosione in alcuni tratti del corso del Reno nella zona collinare appenninica e preappenninica in Provincia di Bologna, sulla base degli elementi acquisiti anche dai competenti uffici territoriali, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto è necessario rilevare che le sponde del Reno in vari tratti, anche più a valle di quelli segnalati, presentano localizzate situazioni di erosione. Per quanto attiene alle problematiche ingeneratesi a seguito degli eventi di febbraio e marzo 2016, il Consiglio dei ministri ha provveduto a contemplare tali aree nell'ambito del provvedimento di delibera di riconoscimento dello stato di emergenza del 10 maggio ultimo scorso richiesto dalla Regione Emilia-Romagna. Con tale delibera sono stati assegnati 9.200.000 euro quale contributo straordinario per l'attuazione dei primi interventi. Tuttavia, ferma restando la possibilità di specifici e localizzati interventi urgenti a tutela di aree con elevati livelli di rischio idraulico che il commissario delegato, Presidente della Regione, potrà valutare nella predisposizione del piano degli interventi, è da evidenziare che, per quanto riguarda sia il Reno che, in modo abbastanza generalizzato, il reticolo idrografico dei territori della Provincia di Bologna, saranno fondamentali gli interventi di complessiva sistemazione idraulica che nei prossimi anni si renderanno possibili nell'ambito degli strumenti di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo per la mitigazione del rischio, che vedono impegnati la Presidenza del Consiglio del territorio e del mare e la Regione Emilia-Romagna. Tale complessiva programmazione di difesa del suolo appare la più idonea a garantire che gli interventi che vanno a modificare velocità e direzione della corrente e le associate condizioni di trasporto solido sempre ben inquadrati e opportunamente verificati nell'ambito del bacino di riferimento; ciò al fine di garantire il controllo e, ove possibile, la riduzione a livelli compatibili del rischio idraulico alla scala di bacino. Per quanto riguarda, nello specifico, la morfologia e il tracciato dell'asta del fiume Reno nel tratto montano da Bocca Nord, in sponda destra, a Borgata Molinaccio, in sponda sinistra, nei Comuni di Castel di Casio e Gaggio Montano, frazione Marano di Gaggio, si fa presente che essi non hanno subito modificazioni rilevanti nell'ultima decade e che i fenomeni erosivi indicati sono tipici di una dinamica fluviale naturale non particolarmente critica. l'alveo inciso del corso d'acqua, definito dalle sponde, è delimitato dalla presenza di vegetazione arbustiva e arborea, boschi in destra e sinistra idraulica, limitate aree a seminativo e a prato stabile e da pochi fabbricati sparsi, comunque sufficientemente lontani dalle sponde stesse e non direttamente interessati dall'erosione. In ogni caso, il tratto è stato particolarmente monitorato nel tempo, in quanto interessato dai lavori di realizzazione della nuova strada statale Porrettana, oggi terminati. Tale monitoraggio ha consentito di determinare che i lavori stessi non hanno comportato significative variazioni al tracciato e alle caratteristiche fluviali, rimaste pressoché inalterate nel tempo, salvo in punti localizzati. Nel tratto sono presenti alcuni tralicci ENEL, regolarmente concessionati. Risulta comunque a carico del gestore l'eventuale protezione dei tralicci stessi qualora, per motivi idraulici, possano venirsi a modificare le condizioni di sicurezza degli stessi. Analogamente, per quanto riguarda il metanodotto, la risoluzione di eventuali problematiche sono anch'esse a carico del gestore. Al riguardo, sulla base delle informazioni in possesso dell'ente competente, non si rileva, allo stato attuale, la necessità di procedere a interventi diffusi di messa in sicurezza sull'intero tratto, che potrebbero anzi comportare un'alterazione dell'equilibrio dinamico dell'asta. In ultimo, si evidenza che il competente ufficio della Regione Emilia-Romagna ha confermato che si provvederà a fare ulteriori sopralluoghi nell'area, anche in accordo con i Comuni interessati, finalizzati a verificare in dettaglio eventuali erosioni localizzate e valutando le eventuali possibili azioni. Per quanto riguarda le misure da adottare finalizzate a contenere il fenomeno della graduale erosione, gli enti territoriali competenti per l'ambito di riferimento della zona interessata, seppur vincolati dagli inevitabili limiti imposti dalle risorse economiche assegnate, e quindi chiamati a valutare attentamente le priorità di intervento, sulla base di valutazioni del rischio riguardanti l'intero territorio di competenza, operano generalmente con la dovuta attenzione, competenza e tempestività.

Sono abbastanza soddisfatta della risposta. Mi premeva portare all'attenzione del Governo il problema dell'erosione del territorio e, nello specifico, della mia zona,

la zona perché abbiamo visto che il fiume Reno è a rischio ingrossamento e pertanto potrebbe danneggiare i terreni agricoli circostanti. Sappiamo che l'agricoltura rappresenta un importante settore economico per la Regione Emilia-Romagna.

con riferimento alle questioni poste dall'interrogante, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue. La normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque

Le citate norme comunitarie, e le norme nazionali di recepimento, definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le autorità competenti per le attività di monitoraggio, definiscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e il controllo di qualità, stabiliscono la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i relativi *standard* di qualità e i valori soglia e le metodiche di analisi. Inoltre, nel gennaio del 2014 è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della direttiva 2009/128/CE. Tale direttiva riguarda solo i prodotti fitosanitari, mentre per i biocidi la Commissione europea sta predisponendo un atto specifico. Il predetto Piano nazionale prevede una serie di azioni, la cui attuazione è demandata in parte alle Regioni e in parte alle amministrazioni centrali competenti (Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute). Con riferimento alle attività di monitoraggio, le Regioni e le Province autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, realizzano il monitoraggio nell'ambito dei programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sottopongono a monitoraggio nei corpi idrici superficiali le sostanze prioritarie e le altre sostanze che non consentono il conseguimento del buono stato entro le date fissate e trasmettono i risultati all'ISPRA, che li elabora e valuta. Si sottolinea che, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli *standard* di qualità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee non vengano rispettati, è necessario attuare le misure di ripristino, che devono far parte dei cosiddetti «programmi di misure» dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE. Allo scopo di valutare l'efficacia delle azioni previste dal Piano di azione nazionale, sono stati definiti con decreto del 15 luglio 2015 alcuni indicatori per valutare il grado di attuazione e l'efficacia delle misure previste. Tali indicatori si basano sui dati di monitoraggio forniti dalle Regioni ed elaborati annualmente dall'ISPRA. L'ISPRA realizza il Rapporto nazionale pesticidi nelle acque nel rispetto dei compiti stabiliti dal Piano. Il Rapporto contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee, le cui finalità sono quelle di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei pesticidi, non previsti nella fase di autorizzazione e non adeguatamente controllati nella fase di utilizzo. L'istituto fornisce, altresì, gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e l'esecuzione del monitoraggio. Per quanto riguarda le sostanze da considerare nel monitoraggio, la normativa acque indica come criterio generale quello di esplorare tutte le potenziali fonti di contaminazione presenti sul territorio, che potrebbero avere un impatto sulle acque. Nei fatti, però, la normativa esplicita solo un certo numero di pesticidi. Pertanto, per avere un quadro completo della possibile contaminazione da pesticidi, l'ISPRA è impegnata nell'attività di indirizzo, in particolare per fornire criteri ed elenchi di sostanze prioritarie da inserire nel monitoraggio. I documenti di indirizzo prodotti sono sul sito *web* dell'istituto ISPRA. L'ISPRA è, altresì, impegnata da anni a fornire tutte le informazioni necessarie alla messa in atto di un monitoraggio rappresentativo dei pesticidi, anche attraverso l'armonizzazione delle attività regionali, fornendo in tal modo un'informazione adeguata ai cittadini sullo stato della contaminazione ambientale da pesticidi, ma anche alle autorità competenti in materia per l'assunzione, quando necessario, di decisioni in materia di gestione del rischio. Al riguardo, tuttavia, si riscontrano ritardi, in particolare in alcune Regioni del Sud Italia. Anche grazie all'azione di coordinamento di Ministero dell'ambiente e alla collaborazione di ISPRA con le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, si sta cercando di recuperare tali ritardi.

Con riferimento all'aggiornamento dei parametri, delle metodologie e dei valori utilizzati per il controllo e il monitoraggio delle acque, a livello nazionale si opera coerentemente alle norme vigenti a livello comunitario. Le stesse norme comunitarie prevedono infatti un riesame e un adeguamento periodico dei parametri e delle metodologie, ove necessario. La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ad esempio, prevede un riesame e una eventuale revisione e integrazione della lista delle sostanze di priorità ogni quattro anni. L'Italia, oltre a partecipare a tale attività, secondo i meccanismi puntualmente definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, assicura il proprio contributo, anche attraverso gli istituti di ricerca nazionali, ai tavoli di lavoro comunitari che preparano a livello tecnico le attività di riesame e revisione, quali ad esempio il gruppo di lavoro "sostanze chimiche" che opera nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque. Anche riguardo alle acque sotterranee, la direttiva 2006/118/CE prevede un riesame periodico e un'integrazione dei parametri sottoposti a controllo. In proposito, il Ministero dell'ambiente ha proceduto a predisporre la proposta di recepimento della direttiva 80/2014/UE, che tra l'altro introduce un nuovo parametro da sottoporre a monitoraggio. Nel provvedimento di recepimento, il Ministero dell'ambiente ha proposto l'introduzione di valori soglia nelle acque sotterranee per 5 composti perfluoroalchilici, sulla base della constatata diffusione a livello nazionale di tale sostanza nelle acque. Le autorità competenti, cui la normativa assegna i compiti di monitoraggio e controllo dei corpi idrici, dispongono pertanto degli strumenti normativi e tecnici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici, secondo i criteri e i metodi definiti dalla normativa europea. Per quanto concerne la disciplina del recupero dei fanghi, occorre rilevare inoltre che la direttiva 86/278/CEE in vigore, dopo quasi trent'anni dalla sua adozione, appare superata, in quanto ad oggi vengono utilizzate sostanze chimiche nuove rispetto al passato. Per questo motivo alcuni Stati membri ed anche alcune Regioni italiane hanno emanato ed implementato misure più restrittive per quanto riguarda i valori limite dei metalli pesanti, così come per alcuni contaminanti per i quali la direttiva non prevedeva limiti. Si assiste dunque ad un'applicazione non omogenea sul territorio nazionale ed europeo della disciplina del recupero dei fanghi in agricoltura, con limiti e requisiti diversi da Regione a Regione. Alla luce di ciò si fa presente che la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel passato (2009-2011) ha già intrapreso attività di aggiornamento degli allegati del decreto legislativo di recepimento della predetta direttiva, che richiedono comunque un necessario coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti. Peraltro, per quanto riguarda le azioni di tutela dell'ambiente acquatico, sono state stabilite, con decreto ministeriale del 10 marzo 2015, linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Tali linee guida prevedono diciotto possibili misure di mitigazione del rischio, che possono essere adottate in relazione a diversi obiettivi di protezione e la cui scelta è demandata alle Regioni e alle Province autonome. I risultati derivanti dall'applicazione di tali misure in termini di minore impatto ambientale potrebbero essere valutati e apprezzati già a partire dal monitoraggio del 2017. Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, anche al fine di superare le eventuali criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina.

superare le criticità legate alla vetustà della direttiva europea. Speriamo che ci arrivi proprio dall'Unione europea una revisione più organica. Credo che tutto questo si inquadri in una situazione di grave timore per la salute dei cittadini, come abbiamo visto anche in alcune Regioni, in particolare del Nord. Sappiamo che sul tema dei PFAS c'è una criticità molto forte, attualmente individuata in Veneto, ma non sappiamo

il senatore Scalia chiede l'avviso del Ministero in merito al progetto del Comune di Frosinone per la riqualificazione di piazza Risorgimento. Vorrei opportunamente evidenziare che i lavori di riqualificazione di piazza Risorgimento in Frosinone fanno parte del piano di recupero dell'ex Casa circondariale, che ha visto l'avvio dell'*iter* amministrativo nei primi anni Duemila. Da allora il progetto è stato oggetto di diversi aggiornamenti che hanno ottenuto la prevista autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del codice. L'ultimo aggiornamento progettuale in ordine di tempo è stato approvato nell'aprile del 2011. Da allora non è stata comunicata alcuna data di inizio lavori, condizione necessaria per dare avvio ai lavori, così come disposto nell'autorizzazione. Nel maggio del 2015, è pervenuto alla competente Soprintendenza per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo un esposto anonimo che denunciava «la cementificazione di piazza Risorgimento a Frosinone, con affossamento della fontana ivi presente di 30-40 centimetri e la realizzazione attorno al monumento di Vittorio Emanuele II di muri, muretti e scalette». A seguito di tale esposto, il Soprintendente incaricava il funzionario di zona di verificare la fondatezza di quanto denunciato nell'esposto. Nel sopralluogo effettuato dall'architetto incaricato emergeva che erano in effetti in corso di esecuzione lavori di sistemazione dell'area difformi dalle previsioni progettuali approvate dalla Soprintendenza nell'aprile del 2011. La stessa Soprintendenza richiedeva urgenti chiarimenti all'amministrazione comunale circa i lavori in esecuzione e contestualmente informava doverosamente la procura della Repubblica, il comando di polizia municipale, il comando carabinieri di Frosinone e la Regione Lazio per gli eventuali e autonomi accertamenti. L'amministrazione civica, in riscontro della richiesta di chiarimenti, segnalava, nel luglio del 2015, che - cito testualmente - «erano in corso di esecuzione lavori di sistemazione dell'area identificabile come piazza Risorgimento, consistenti nella pavimentazione di spazi pedonali in conformità al progetto autorizzato dalla Soprintendenza, posticipando a successivo intervento per giustificati motivi di costo, la analoga pavimentazione delle zone destinate alla percorrenza dei veicoli, che saranno mantenute in asfalto. Nell'intervento sono state inoltre inserite tutte le misure idonee al superamento delle barriere architettoniche in conformità delle vigenti disposizioni di legge. Gli adempimenti di cui sopra, che rappresentano che rappresentano necessario sviluppo in fase esecutiva del richiamato progetto approvato dalla Soprintendenza (...) non sono stati oggetto di formalizzazione per mero disguido» - ribadisco e sottolineo: per mero disguido «Con plico a parte si inoltra il progetto adeguato per il seguito di competenza». Fine della citazione. ordinava la rimessa in pristino della condizione della piazza antecedente alle opere non autorizzate per il fatto che i nuovi interventi incidevano negativamente sul contesto storicizzato e tutelato. Con lo stesso provvedimento imponeva altresì il pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per l'omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del codice dei beni culturali per le opere realizzate (con marcato stravolgimento del progetto allora approvato). Il Comune impugnava il provvedimento di rimessa in pristino della soprintendenza e la questione è ancora pendente avanti il TAR Lazio - sezione staccata di Latina. Permettetemi qui di sottolineare, proprio dalla successione dei fatti, che è l'amministrazione civica ad aver omesso, nella fase autorizzatoria e poi esecutiva dell'opera pubblica, la necessaria interlocuzione con questo Ministero, impedendo impedendo alla Soprintendenza di svolgere quelle funzioni di alta sorveglianza cui essa è preposta e che avrebbero impedito quanto accaduto. Inoltre le varianti di opere pubbliche interessanti beni culturali, al pari dei progetti, vanno assoggettate preventivamente alla valutazione della Soprintendenza. Diversamente, ad opera conclusa o quasi, le opere abusivamente realizzate sono assoggettate in ogni caso alle sanzioni previste dal codice. Nella sostanza tutte le lavorazioni eseguite non appaiono giustificate dalla condivisa esigenza di abbattere le barriere architettoniche. Piazza Risorgimento, nella configurazione *ante* opera, presentava infatti un'area pubblica deputata alla sosta/incontro, tagliata in due dalla carreggiata destinata al traffico veicolare che determina due distinte aree pedonali, una a valle dove è presente una fontana e una a monte con il monumento a Vittorio Emanuele II. L'area più a valle dove insiste la fontana e diverse alberature era caratterizzata in origine da un lieve dislivello. Con i lavori in questione si è artificiosamente livellato il terreno e rialzata la quota di calpestio attorno alla fontana, determinando l'affossamento della stessa oltre all'amplificazione delle problematiche di accessibilità per i diversamente abili, alle quali si è posto rimedio con la realizzazione di due lunghe rampe inclinate delimitate da muretti in cemento armato. Nella fattispecie si ritiene che i problemi di accessibilità potessero essere risolti più agevolmente, e devo dire con minore enfasi, mantenendo le quote di calpestio originali. In buona sostanza con il rialzo delle quote si sono create barriere architettoniche per poi eliminarle. Nell'area più a monte dove è collocato il monumento e dove la pendenza diventa più accentuata, i lavori eseguiti hanno determinato un radicale cambiamento del previsto schema compositivo e di gestione degli spazi destinati alla sosta e delle aree lasciate a verde. È proprio tale radicale cambiamento della piazza che doveva essere preventivamente autorizzato. Concludo precisando che il Comune di Frosinone, di recente, ha trasmesso alla Soprintendenza alcuni nuovi progetti di rimessa in pristino della piazza Risorgimento e la Soprintendenza si è espressa in linea di massima favorevole ad una delle proposte ed è in attesa di ricevere - speriamo tutti in tempi brevi - un progetto di maggior dettaglio che coniughi il ripristino delle quote originarie con le previsioni progettuali di riqualificazione già approvate nell'aprile del 2011.

perché «la sistemazione proposta appare eccessivamente subordinata alle esigenze di accessibilità per i diversamente abili». È nota la normativa che impone di adeguare i progetti all'eliminazione delle barriere architettoniche e mi risulta dalla scheda del Comune che poi mi ha trasmesso che l'unica ipotesi progettuale che viene condivisa dalla Soprintendenza è il ripristino della situazione *quo ante* che il Comune ritiene non praticabile. Se possibile inviterei a un ulteriore approfondimento, perché proprio nel giudizio a cui lei faceva riferimento c'è stata una fase cautelare e il Consiglio di Stato ha invitato il TAR a entrare nel merito celermente e ad accertare se ci sia l'interesse culturale perché il bene di cui si parla è una fontana della Cassa del Mezzogiorno di meno di settant'anni, rispetto alla quale non c'è evidenza che ci sia stata la verifica dell'interesse culturale da parte del Ministero e da parte della Soprintendenza, come avrebbe dovuto essere

dell'opera di urbanizzazione che era tenuto a fare il privato. Qui c'è stato - come ha ricordato il Sottosegretario - un piano di recupero di iniziativa privata che è stato realizzato per la parte di interesse privata, ma non è stata organizzata l'opera di urbanizzazione e la sistemazione della piazza, cui sta provvedendo il Comune con la polizza fideiussoria che ha escusso in danno al privato. Per cui quel piano è già stato realizzato, la piazza è già stata stravolta e l'immobile è già stato realizzato. Ora va risistemata la piazza e va resa percorribile, perché da diversi da diversi anni è impraticabile. Quindi, l'urgenza è di consentire una sistemazione che sia coerente con la normativa che impone l'eliminazione delle barriere architettoniche. Se questo disturba il senso estetico della Soprintendenza, accertiamo se quest'ultima ha su quel bene un